Gentile Presidente, informo la Signoria Vostra che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, sentito il Consiglio dei ministri, ha nominato i seguenti Sottosegretari di Stato:

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il calendario dei lavori fino al 9 marzo. In relazione all'*iter* in Commissione del decreto-legge recante ulteriori per le elezioni 2021, già all'ordine del giorno di oggi, la discussione del provvedimento avrà inizio nella seduta di domani, a partire dalle ore 10. Giovedì 4 marzo, alle ore 10, sarà discusso dalla sede redigente il disegno di legge sulla dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano. Alle ore 15 avrà luogo il *question time*, con la presenza dei Ministri delle politiche agricole, per le politiche giovanili e per i beni culturali. La settimana dall'8 al 12 marzo sarà prevalentemente riservata ai lavori delle Commissioni, con particolare riguardo alle audizioni sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'Assemblea si riunirà nella giornata di martedì 9 marzo, alle ore 16,30, per la discussione del decreto-legge sul funzionamento del CONI. Alle ore 15 di martedì 9 marzo è convocata la Conferenza dei Capigruppo per definire il prosieguo dei lavori. La Presidenza ha nuovamente richiamato l'attenzione dei Capigruppo circa i criteri di redazione degli atti di sindacato ispettivo, basati sulla rigorosa applicazione delle norme regolamentari, secondo le direttive già comunicate l'11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

Non lo ha fatto per un capriccio, per il gusto di essere contro tutto e contro tutti, ma dopo aver tentato lungamente, nel corso di tutta la Conferenza dei Capigruppo, di trovare un accordo onorevole per tutti. Invece, l'atteggiamento, purtroppo, non è stato di questo genere. Noi non siamo entrati in quella riunione con alcun pregiudizio nei confronti della maggioranza. Abbiamo ascoltato le ragioni del Governo, che sono ragioni che hanno una loro forza. Noi riconosciamo, infatti, il diritto-dovere del Governo di fare approvare i propri provvedimenti,

proprie ragioni, poter portare all'attenzione del Governo e dei colleghi le motivazioni di chi non ha condiviso le scelte di maggioranza. È un ruolo altrettanto importante di quello di chi governa.

che i diritti minimi della minoranza vengano calpestati né in Assemblea, né in Commissione, né nel corso delle riunioni dei Capigruppo. Voglio dirlo in maniera molto chiara e molto netta; se qualcuno si attende che la nostra ragionevolezza sia confondibile con altri atteggiamenti di totale genuflessione nei confronti della maggioranza ha sbagliato indirizzo ed è meglio che se lo metta chiaro in testa Noi ricorreremo a tutti gli strumenti che il Regolamento consente per difendere le nostre ragioni, che non sono quelle di Fratelli d'Italia, ma quelle dell'opposizione che deve essere considerata per il merito che ha. Esprimeremo pertanto un voto contrario sul calendario e, se l'atteggiamento della maggioranza sarà di questo stampo, credo che sarà contrario anche nelle prossime occasioni. finestra"). Senatore Ciriani, la Presidenza ha preso buona nota delle sue argomentazioni.

DRAGO *(Misto)*. Signor Presidente, colleghi, vorrei porre alla vostra attenzione una questione che riguarda un cospicuo numero di docenti che oltre ad essere esiliati, sono diventati anche invisibili il vaccino degli insegnanti. Si stanno verificando infatti situazioni paradossali in quanto i docenti titolari di posto in una Regione diversa dalla propria residenza non riescono ad accedere al servizio di prenotazione vaccinale in quanto il sistema non li riconosce né nella Provincia di residenza, né in quella di titolarità. Su questo ci si dovrebbe impegnare celermente a dipanare la matassa dipanare la matassa in cui sono ingabbiati e avvolti, per non vanificare gli sforzi che si stanno facendo per vaccinare il personale scolastico. Colgo l'occasione, inoltre, per rammentare che circa 15.000 di questi sono in attesa di mobilità, come previsto da numerose sentenze.

cento iniziale dell'anno 2019-2020, si è giunti ad un 25 per cento per l'anno 2021, a causa del contratto integrativo vigente, un numero decisamente basso che in questi tempi di pandemia non riesce a garantire, se non a pochissimi,

Signor Presidente, la nave Brod Mira Galeb, residenza marittima del maresciallo Tito, verrà trasformata, grazie al sostegno di un finanziamento europeo ottenuto dalla Croazia nell'ambito del progetto di valorizzazione turistica dei monumenti rappresentativi del patrimonio industriale di Fiume, in un museo multimediale. L'obiettivo è quello di rendere la nave luogo di attrazione attrazione culturale e turistica della città di Fiume, grazie ad una allocazione di 9,259 milioni di euro. Se è vero che i fondi europei dovrebbero essere elargiti con l'obiettivo di valorizzare un patrimonio la cui preziosità è trasversalmente riconosciuta e mai per alimentare faziosità ideologica, il finanziamento concesso rischia di essere percepito come omaggio al maresciallo Tito, colpevole di uccisioni di massa, oltre che della promozione di una vera e propria pulizia etnica, aggravata da fattore ideologico e dunque come un tentativo di promuovere una lettura della storia che interpreti il comunismo come una fase di opinabile brutalità.

condanna alla detenzione per infrazione alle legge sugli ammassi obbligatori. Gli oppositori del regime sparivano, naturalmente senza lasciare traccia; 12.000 carcerati di Istria e Quarnero furono rieducati con atroci torture fisiche e psicologiche, molti non tornarono a casa. Il marchio più infamante nella storia di Tito parte dai *lager* jugoslavi, detti i campi della morte, che ancora oggi gridano vendetta, lo stesso grido che risuona dal buco nero delle foibe, che continuano a moltiplicarsi. Nei rapporti stilati da uomini dei Servizi speciali della Marina, emergono una cinquantina di pagine corredate da testimonianze agghiaccianti e fotografie inequivocabili, veri e propri campi di concentramento sfuggiti alla ribalta mediatica dei più conosciuti campi tedeschi. Il dittatore Tito ha utilizzato lo strumento del terrore per tenere uniti i popoli di variegate razze e religioni. A lui va addebitato, oltre ogni ragionevole dubbio, l'atroce appellativo di inventore della pulizia etnica. È per questo che il sostegno dato da parte dell'Unione europea all'iniziativa di restauro rischia di apparire contrario a quanto affermato dal Parlamento europeo all'interno della risoluzione del 19 settembre 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa, se i crimini titini e la politica di repressione antidemocratica non venissero inquadrati all'interno del percorso museale in cui l'opera intende inserirsi. In tal senso auspico che il Governo italiano si faccia portavoce presso la Commissione europea e presso il Governo croato affinché questi elementi di verità... PRESIDENTE. Le ho dato qualche minuto in più per l'interruzione e anche per l'importanza del tema che lei ha trattato.

Invece di autoassolversi in ridicole autointerviste, Renzi dovrebbe vergognarsi, scusarsi pubblicamente e dimettersi immediatamente dal consiglio della fondazione saudita «Future investment initiative institute», dalla quale percepisce 80.000 euro annui. Il suo amico principe saudita, bin Salman, da Renzi definito un campione del nuovo Rinascimento mediorientale, un sovrano moderno e illuminato, che tutto il mondo arabo dovrebbe prendere come esempio, è stato ufficialmente riconosciuto dagli Stati Uniti responsabile del barbaro assassinio del giornalista Jamal Khashoggi, ammazzato e letteralmente fatto a pezzi per aver criticato la sua monarchia: roba degna del più buio Medioevo, altro che Rinascimento! Come del resto i 3.000 bambini yemeniti trucidati dai selvaggi bombardamenti aerei sauditi su villaggi, mercati, moschee, scuole e ospedali, e gli 85.000 bambini morti a causa della carestia provocata in Yemen dall'assedio militare saudita. La differenza di spessore umano, prima che politico, tra noi e Renzi, sapete qual è? Ve lo dico io: negli stessi giorni in cui Renzi, in piena pandemia e in piena crisi di Governo, da lui stesso provocata, se ne andava in Arabia Saudita, dietro lauto compenso, a tessere le lodi di un regime violento, il governo di Giuseppe Conte e la Farnesina guidata da Luigi Di Maio bloccavano la vendita di armi verso quello stesso regime. Tra esse le oltre 20.000 bombe prodotte in Italia, che proprio Renzi nel 2016, da presidente del Consiglio, aveva deciso di vendere al suo amico bin Salman, quando i crimini di guerra sauditi in Yemen erano noti già da tempo. Voglio credere non vi sia alcuna correlazione tra il sostegno garantito da Renzi allo sforzo bellico saudita in Yemen e la fruttuosa collaborazione che lo stesso si è poi visto offrire dal capo di quella Nazione. Ritengo comunque doveroso avviare una riflessione sull'opportunità politica ed etica che i parlamentari in carica percepiscano somme di denaro per la loro partecipazione ad associazioni, fondazioni e simili. Per questo valuterò eventuali ulteriori azioni, anche legislative, volte a sanare quella che, a mio avviso, è una questione da affrontare in modo serio. Concludo: purtroppo il collega Renzi, come sovente accade, non è presente in Aula, perché gli avrei voluto dire *vis a vis* che, se ha un minimo di coscienza, dovrebbe interrompere subito i suoi rapporti di collaborazione retribuita con la fondazione saudita e donare gli 80.000 euro che ha percepito ai cinque figli di Khashoggi, oppure ai parenti della famiglia yemenita (padre, madre incinta al quarto mese e quattro bambini), sterminata l'8 ottobre 2016 in un villaggio

Signor Presidente, siamo costantemente sottoposti ad un'emergenza dentro l'emergenza: lo abbiamo detto in diverse circostanze. Ebbene, ritengo altresì che sia davvero un'emergenza affrontare l'ipocrisia del nostro Paese, che trova supporto e conforto in certo giornalismo, avvalorato dalla presenza di un senatore della Repubblica: Matteo Renzi. *(Commenti)*. Questo mio intervento nasce dall'esigenza di porre i riflettori su quanto accaduto qualche giorno fa,

tratta del giornalista, oppositore del regime di Riad, che ha palesato di mettersi contro le scelte del principe Moḥammad bin Salman, assassinato il 2 ottobre 2018. Questo caso, che ha coinvolto proprio il principe saudita bin Salman, pretende un'assunzione di responsabilità e di serietà, sia da parte della narrazione mediatica sul caso, sia da parte del senatore Renzi. Dunque, ripercorriamo un po' quello che è accaduto: il senatore in questione innesca la crisi in Italia, in un momento storico più che mai fragile, complesso e complicato, facendo dimettere due Ministri e un Sottosegretario. Egli, però, in piena crisi, da conferenziere ben pagato, si reca in Arabia saudita, rientra in Italia per le consultazioni con il presidente Mattarella e, nel momento dell'informativa televisiva, trasforma abilmente quel breve momento di coinvolgimento dei nostri

giorno dell'assassinio di Khashoggi, il senatore della Repubblica Renzi si sia recato in Arabia saudita. Certamente il ruolo da conferenziere lo ha ottenuto proprio grazie alla politica e dalla politica dovrebbe appunto dimettersi, data la gravità di questi fatti, fatti, che si riscontra anche nella becera complicità della stampa, dal silenzio comunque assordante. Auspicando dunque che il senatore Renzi possa dimettersi quanto prima, gli ricordo le sue stesse parole, tutto la settimana dopo la fine della crisi di Governo. Senatore, aspettiamo con ansia, e colgo l'occasione per ringraziare il nostro ministro degli affari esteri, Luigi Di Maio, per l'impegno profuso.